verificare. Il Senato è in numero legale.

il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 8 maggio 2009 Onorevole Presidente, informo la S. V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato Ministro senza portafoglio l'on. Michela Vittoria BRAMBILLA, la quale cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cordialmente *F.to* Silvio Berlusconi»

Onorevoli colleghi, la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì, si è spento nella sua casa di Genova don Gianni Baget Bozzo. ottantaquattro anni fa, sul finire della guerra entrò in contatto, durante gli studi universitari, con il movimento clandestino della Democrazia cristiana genovese, guidato da Paolo Emilio Taviani, e divenne rapidamente responsabile del movimento giovanile democristiano della sua città, partecipando anche all'insurrezione di Genova contro le truppe di occupazione naziste. Dopo la Liberazione, avvicinatosi alle posizioni di Giuseppe Dossetti, iniziò a ricoprire incarichi di responsabilità all'interno della Democrazia Cristiana: il dibattito interno al partito sull'opportunità di avviare la collaborazione di governo con il Partito socialista, acuitosi nel corso della III legislatura con la tumultuosa vicenda del Governo Tambroni, condurrà Baget Bozzo verso posizioni critiche nei confronti della maggioranza democristiana. I suoi scritti di quel periodo manifestano una straordinaria capacità di analisi delle esigenze e dei limiti della democrazia italiana, ed anticipano temi e questioni che diverranno dominanti, nel dibattito pubblico, soltanto molti anni dopo, come la critica alla partitocrazia e le riflessioni sull'opportunità di riformare in senso presidenziale la nostra forma di Governo. Nel frattempo, però, alle difficoltà della vita politica attiva si accompagnò una forte esperienza mistica che condusse Baget Bozzo a concentrare la sue energie di intellettuale sulle grandi questioni teologiche ed ecclesiali sollevate dal Concilio Vaticano II, nella convinzione che il futuro della Chiesa cattolica e gli orizzonti della civiltà umana, in primo luogo di quella italiana ed europea, fossero tra loro intimamente legati. Quell'esperienza mistica porterà questo raffinato intellettuale e commentatore politico a rispondere anche, finalmente, alla sua vocazione giovanile, ricevendo l'ordinazione sacerdotale dalle mani dell'arcivescovo Giuseppe Siri nel novembre del 1969. Un altro evento traumatico della vita politica italiana, quale il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro nel 1978, contribuì ad allontanare ulteriormente don Gianni Baget Bozzo, favorevole alla trattativa con le Brigate rosse, dalla linea del suo partito, e ad avvicinarlo alle posizioni espresse dal Partito Socialista, guidato da Bettino Craxi. Questo processo di graduale distacco dalla Democrazia Cristiana e di convergenza nei confronti della nuova formazione politica culminò nel 1984, con l'accettazione della candidatura, nelle liste socialiste, alla carica di parlamentare europeo, e con la successiva elezione, confermata anche nella legislatura successiva, fino al 1994. Questa scelta, motivata dalla volontà di offrire un segnale di opposizione al principio dell'unità politica dei cattolici, considerato non più adeguato alle istanze di modernizzazione della politica italiana, gli comportò la sanzione canonica della sospensione dall'esercizio delle funzioni sacerdotali, da lui vissuta con grande dolore, proprio a causa dei suo radicato sentimento di attaccamento alla Chiesa e al suo Arcivescovo. Dopo il 1994, terminata l'esperienza parlamentare, Baget Bozzo tornò alla sua occupazione prediletta di saggista e commentatore politico. Le sue prese di posizione sulla politica italiana dell'ultimo quindicennio, talora assai controverse, confermavano la sua natura di pensatore libero e indipendente, mai preoccupato di discostarsi dall'opinione dominante, anzi sempre pronto, anche attraverso la provocazione intellettuale, a stimolare il dibattito e la riflessione critica dei suoi interlocutori. Con don Gianni Baget Bozzo ci si poteva trovare in sintonia o in contrasto, ma certamente nei suoi confronti non si rischiava di provare indifferenza. Penso di rendergli un omaggio non convenzionale ricordando che proprio l'allora cardinale Ratzinger era il 2002 - sebbene non condividesse pienamente le sue tesi sul cristianesimo scisso dall'idea di religione, lo accostò a Romano Guardini per la distinzione tra fede e religione, così centrale per la teologia e la filosofia delle religioni. A don Giovanni Baget Bozzo, a questa significativa figura di religioso, di intellettuale, di politico, va il nostro commosso ricordo.

la figura di Gianni Baget Bozzo è stata assai significativa sia per la biografia personale, assolutamente anomala e desueta, sia per la vicenda politica, che ha intrecciato la vita sacerdotale. La complessa infanzia e le difficoltà dei primi anni di vita lo hanno forgiato ed hanno permesso alla sua intelligenza fuori dal comune di dedicarsi agli studi ed a quella scrittura che lo rendeva profondo polemista e coraggioso protagonista della vita politica italiana. sua fu una vocazione matura e adulta; divenne prete dopo i quarant'anni, in quella Genova dove fu apprezzato dall'autorevole e rigoroso cardinale Siri, con il quale non mancavano contrasti anche forti. Ricordarlo oggi significa richiamare tutta la sua ricca pubblicistica, dove, nei saggi e negli articoli, sposava le analisi acute e intuitive con il gusto per la parola audace che suscitava scandalo. Ma scandalosa, in senso etimologico, fu la sua vita politica, prima come consigliere e amico di Bettino Craxi, che lo volle europarlamentare, incarico che accettò e che gli costò la sospensione dall'esercizio sacerdotale; ne soffrì, ma non esitò a buttarsi nell'avventura di Forza Italia, accanto a Silvio Berlusconi, del quale è stato sino all'ultimo uno dei consiglieri più ascoltati. Verso il movimento della Lega Nord ebbe attenzione e condivisione di alcuni temi fondamentali, soprattutto quelli legati alle politiche identitarie e alla dignità dei popoli. Il suo liberalismo cattolico Il suo liberalismo cattolico non fu mai dogmatico, tanto meno chiuso, ma piuttosto aperto alle novità e alle trasformazioni. Nell'ora dell'addio siamo certi che il suo pensiero possa diventare prezioso patrimonio per gli studi e per quella politica che era la sua autentica passione.

nella giornata di ieri la città di Genova e la chiesa genovese hanno salutato per l'ultima volta don Gianni Baget Bozzo. Noi lo ricordiamo oggi in questa sede perché egli appartiene alla storia politica del nostro Paese. Figlio della terra ligure, egli ha attraversato la storia democratica dell'Italia della seconda metà del Novecento e fino ad oggi con intelligenza e passione, non come un osservatore distaccato, ma come un intellettuale partecipe degli stessi processi storici e politici che acutamente indagava. Prese parte, diventò e fu di parte, prima nella Democrazia Cristiana, poi nel Partito Socialista, in Forza Italia e infine nel Popolo della Libertà. Fu un protagonista originale e creativo, non senza accenti polemici nel dibattito pubblico e nella vita politica. Fu protagonista nel Parlamento europeo europeo e in quelle forme indispensabili all'agire politico che sono l'elaborazione delle idee, l'analisi critica, il suggerimento, l'interlocuzione con il leader, la formazione dei giovani e dei militanti, la divulgazione della cultura politica, la testimonianza generosa. Intellettuale, politico, sacerdote, il suo impegno e il suo coinvolgimento furono totali, senza limiti e senza riserve. A suo modo visse intensamente il suo rapporto con la fede e con la storia, che plasmò la sua vita. Indagò la cristianità, da Costantino al Concilio Vaticano II e sulla frontiera tra Chiesa e mondo, fra cristianesimo e modernità; sviluppò la sua ricerca con libertà e scelte non di rado sorprendenti. Si tuffò poco più che ventenne nel crogiuolo delle idee, degli studi, del dibattito del secondo dopoguerra, aderendo con Dossetti ed altri all'avventura di «Cronache sociali», uno stuolo di giovani, intellettuali e politici, che pensavano e discutevano di economia, di Stato sociale, di partiti, di sindacati, della ricostruzione materiale, culturale e politica del Paese, della politica estera. Portavano in Italia il dibattito internazionale, mettevano le fondamenta della nuova Italia. Mi domando quanto deve essere sembrata lontana, forse, a Baget Bozzo quella stagione, se confrontata con i nostri tempi, con il livello dell'attuale dibattito pubblico del nostro Paese. A me pare che egli sia rimasto coerente con il bisogno di una ricerca più ampia e più profonda, sempre, rispetto alla superficie delle cose e alla loro contingenza. Negli anni Sessanta, sceglie con la rivista "Renovatio" la nostalgia della Chiesa preconciliare e successivamente osteggia il compromesso storico, sceglie Craxi prima e Berlusconi poi, investendo su di essi. È un protagonista entusiasta. Un'intera stagione politica italiana, quella che tuttora viviamo, lo vede protagonista. Noi sappiamo che molte cose ci hanno diviso da lui, nelle scelte intellettuali, nelle scelte religiose, nelle scelte politiche, ma sappiamo anche che la storia politica del nostro Paese ci ha fatto camminare insieme, ed è questo che continua oggi ad interrogarci. Quando muore un protagonista come Baget Bozzo, non si illumina una sponda sola del fiume, si illumina tutto il percorso, il nostro percorso nazionale, i decenni che abbiamo attraversato. La morte parla sempre con la forza che viene dal superamento del limite, dalla distanza, e la sua voce parla anche del significato delle cose che sono consegnate ormai alla storia. Ci costringe a pensarci, a pensare come siamo stati e perché, a quello che siamo diventati gli uni e gli altri, gli uni insieme agli altri, gli uni responsabili anche degli altri, in questi ultimi 20-30 anni.

E di fronte a lui e insieme con lui, il confronto vero era tra coloro che vollero unire, nell'Ulivo prima e nel PD poi, la cultura cattolico-democratica-liberale di sinistra e chi, come Baget Bozzo, vi si opponeva legittimamente e tenacemente, con consapevole riflessione culturale e indomita volontà politica; tra chi indicava una via per l'innovazione e la modernizzazione dell'Italia e chi ne indicava un'altra, ma entrambe si riconoscevano nel medesimo sistema politico bipolare. A ben vedere, il suo percorso personale svela la coerenza di un disegno e la capacità di inverarlo, anche con creatività, nelle condizioni date dalle contingenze politiche, fino ad entrare nella discussione delle idee, dei comportamenti del mondo multiculturale di oggi, con le sue sfide, da quelle date dalle conquiste tecnico‑scientifiche a quelle date da una convivenza tra i diversi. Un disegno, quello perseguito da Gianni Baget Bozzo, a cui non era estranea, e non poteva esserlo, la cultura cattolica, la quale ha variamente ispirato la storia democratica dell'Italia ben oltre l'esperienza della Democrazia cristiana, fino al Partito Democratico e al Popolo della Libertà e ad altre formazioni, con diverse legittime visioni sui fini e sui mezzi. Signor Presidente, con queste consapevolezze il Gruppo del Partito Democratico si unisce oggi al dolore dei familiari di Gianni Baget Bozzo e di quanti lo hanno amato e sentito amico e ispiratore. Sappiamo che mancherà a molti. La sua testimonianza così peculiare lascia un compito a tutti noi, il compito di pensare la politica, di pensarla senza banalità, di sentirla come una grande responsabilità dentro la storia del nostro popolo e del nostro Paese. Qualunque sia la parte in cui militiamo, dobbiamo sapere che costruire una parte significa dare un contributo alla costruzione del tutto, nel confronto aperto che costituisce la vitalità della democrazia. È un compito che non può appartenere ad uno solo o a pochi, ma a tutti. Un partito, un popolo sono un soggetto collettivo. Bisogna che siano un soggetto pensante, consapevole, che guarda avanti, come Baget Bozzo ha testimoniato scegliendo per sé, quasi come una vocazione, questo compito. Ora il suo tempo si è compiuto e si è aperto all'eterno a cui anelava. Ora sta ai confini del tempo, come scrisse in una sua poesia del 1972. Di fronte a noi c'è l'Italia che anche Baget Bozzo ha contribuito a plasmare: dobbiamo augurarci che molti si dedichino alla costruzione del futuro politico dell'Italia con la sua stessa passione culturale, anche se difficilmente con il suo talento. Baget Bozzo se n'è andato nel sonno, alla vigilia del 9 maggio, la giornata dedicata all'Europa, a quell'Europa in cui egli ha creduto. Il 9 maggio 1950 Robert Schuman indicò nella sua storica dichiarazione il sogno nuovo che si apriva davanti agli europei dopo le rovine materiali e morali del conflitto mondiale. In quegli stessi anni - possiamo dire in quegli stessi giorni se andiamo a rileggere «Cronache sociali» - Baget Bozzo vide bene la necessità e la prospettiva del sogno europeo. Forse è lì, cari colleghi, la speranza del futuro che ci unisce, della nuova storia che dobbiamo costruire con la stessa passione culturale e politica che ha testimoniato con la sua vita anche per noi Gianni Baget Bozzo. Signor Presidente, colleghi senatori, se si provasse a mettere in fila le diverse esperienze attraverso le quali la passione politica di Gianni Baget Bozzo si è sviluppata dagli anni Quaranta fino ai giorni nostri, e si ricostruisse questo percorso prescindendo dall'afflato e dalla generosità dell'uomo che lo ha interpretato per oltre mezzo secolo, sembrerebbe quasi di trovarsi di fronte ad un personaggio in cerca d'autore. Ma se si rilegge la storia d'Italia del secondo dopoguerra con gli occhi di don Gianni, se ci si immedesima in questo appassionato pensatore innamorato della libertà, si comprende come le varie tappe della sua vicenda umana siano state, in realtà, momenti di una lettura unitaria e coerente, che di volta in volta ha sperimentato le forme empiricamente più adeguate per farsi politica. Da storico acuto qual era, don Gianni avrebbe tratto grande gusto nell'analizzare la sua vivace biografia e avrebbe trovato qualcosa di straordinario nella parabola esistenziale di un uomo che ha veramente combattuto la Resistenza e che, 15 anni dopo, nel pieno dell'egemonia ideologica dell'antifascismo di Stato, ha avuto il coraggio di classificare il fascismo come fenomeno storico, da sottoporre a valutazione oggettiva, al di là delle categorie tutte politiche di fascismo e di antifascismo; che ha imparato da Dossetti e Maritain che si poteva essere moderni e cristiani al tempo stesso. Ma poi, di fronte all'incalzare della secolarizzazione, piuttosto che aderire alla facile via del rigetto della politica, ha scelto di perseguire una strada più ardua, ma anche più ambiziosa: ricercare la sintesi possibile tra i propri ideali e alcuni esiti della modernità. Mentre il suo percorso subisce questa prima evoluzione, dopo aver militato nelle fila della Democrazia Cristiana del dopoguerra, Baget Bozzo scorge nella svolta a sinistra della stessa DC, la consacrazione di quel "pragmatismo acristiano" contro il quale, attraverso una prospettiva in continua evoluzione, avrebbe lottato per il resto dei suoi giorni. Da qui lo guardo interessato all'esperienza gollista, l'avvicinamento a un Tambroni ormai in disgrazia e ad una giovane generazione destinata a trascorrere gli anni Sessanta chiusa in un ghetto. Negli stessi anni, mentre Moro e Scelba lo aiutano a guadagnarsi da vivere, Baget Bozzo matura la scelta del sacerdozio e diventa collaboratore del cardinale Siri. È anche il momento dell'elaborazione culturale sul fronte storiografico: la Democrazia Cristiana, il tradimento della sua "vocazione", l'apertura a sinistra divengono campi di un'analisi impietosa. Ne scaturiscono libri che ancora oggi resistono come capisaldi della storiografia. Finché, negli anni Settanta, è l'avvento della cosiddetta "società radicale" a stuzzicare l'instancabile curiosità intellettuale di don Gianni e a presentargli una nuova sfida. Di fronte a quella che percepisce come la sostituzione del concetto di bisogno al concetto di individuo, Baget Bozzo avverte l'esigenza di un elemento comunitario e sociale e, in questa fase, guarda con interesse persino al Partito Comunista come possibile interlocutore. Il successivo avvicinamento al Partito Socialista Italiano, e in particolare alla figura di Craxi, non è un ripensamento; è piuttosto un'ulteriore e lineare evoluzione del percorso di un intellettuale demiurgo che persegue un suo coerente disegno ideale di fondo e, di volta in volta, individua il contesto e l'opportunità politica che meglio possano favorire la realizzazione del progetto che ha in mente: sottrarre l'Italia alla morsa delle ideologie e consentire al Paese di trovare una strada lungo la quale le ragioni della modernità possano laicamente comporsi con la nostra identità e la nostra tradizione e "l'evento della libertà" possa ritrovare quel nesso indissolubile con "l'evento cristiano", in una prospettiva in fondo erasmiana, nella convinzione che entrambi gli eventi "si fondano sul concetto che l'uomo sia una persona e che la persona possa creare". Baget Bozzo vedeva lo scorrere di un sentimento popolare profondo al di sotto della marea della cultura dominante. Nell'avvento di Silvio Berlusconi sulla scena politica ha individuato l'occasione affinché, attraverso il riconoscimento reciproco tra il popolo e il *leader*, la sfida fosse lanciata e tale sentimento di libertà potesse emergere e trovare rappresentazione. Poche settimane prima di lasciarci, don Gianni ha potuto assistere - seppure a distanza - alla nascita del frutto più maturo del suo intenso percorso esistenziale: quel Popolo della Libertà al quale ha così profondamente contribuito con il consiglio, lo stimolo e la discussione. In una delle sue ultime lettere, poco dopo la fondazione del nuovo partito, già guardava al passo successivo: come fare ad istituzionalizzare quel fatto sconvolgente per il sistema politico italiano rappresentato da un congresso nel quale si erano incontrati sulla destra dello schieramento politico un popolo, una classe dirigente ed un *leader*. «Vedo che andiamo in questa direzione», scriveva don Gianni, «e il morso che la grande crisi purtroppo farà subire al Paese fonda la possibilità politica» della riforma costituzionale. Trarre forza dal momento di difficoltà e cogliere l'opportunità storica di modernizzare le nostre istituzioni: questo è l'ultimo grande compito che don Gianni ci ha lasciato in eredità. Faremo di tutto, don Gianni, per essere all'altezza della tua generosità, della tua passione e della tua speranza! Grazie,

quella di don Gianni Baget Bozzo è una figura di straordinaria ed intensa vivacità intellettuale, politica, civile e morale, all'interno della quale però si coglie con grande facilità - è stato pure ricordato

Don Gianni si è scontrato con il potere politico e anche con una certa visione e lettura della Chiesa cattolica; eppure è stato

di Gianni Baget Bozzo, che appartiene a quella categoria di persone di cui il Paese rischia di scoprire solo troppo tardi o dopo la loro scomparsa lo straordinario contributo che hanno dato

Ebbene, Presidente, ci sono due elementi sui quali il pensiero di Baget Bozzo si è in particolare soffermato nel corso dei suoi scritti e della sua azione politica. Credo che possiamo dire, senza che questo diventi motivo di divisione tra i Gruppi o tra i partiti,

Grazie, fortemente in passato, lui da cattolico, con una certa cultura del partito cattolico e a farlo ritrovare invece più agevolmente nelle file laiche, riformiste, socialiste di Forza Italia e del Popolo della Libertà. Eppure, Presidente, c'è un'altra passione, un impegno politico, intellettuale e civile, nel quale don Baget Bozzo è stato precursore e ha speso tante energie, che non ha trovato ancora compimento. L'auspicio del Governo è che

Signor Presidente, illustrerò il complesso degli emendamenti che gli esponenti del Partito Democratico hanno presentato all'articolo

Ciò detto, il discorso è più politico e più complessivo. Vediamo che il Governo, lo stesso ministro Scajola e anche la ministra Prestigiacomo

parole del Governo - contando anche sul qualificato contributo di professionalità e di esperienze che può giungerci dalle imprese americane. Mi pare alquanto surreale che su un tema così strategico e delicato il Governo avverta la necessità di puntare su professionalità straniere, dimenticando che da tempo i nostri cervelli sono in fuga, cervelli del calibro del premio Nobel Rubbia. Forse però la concezione del Governo non è proprio una dimenticanza, visto che Rubbia è stato costretto ad emigrare in Spagna per continuare la sua ricerca sui reattori di quarta generazione, non di terza, e sul solare termodinamico. Egli ha certamente le idee chiare, cosa che non mi pare questo Governo abbia. Anche in Commissione abbiamo sostenuto che si doveva puntare sulla quarta generazione nel momento in cui si intraprendeva questa strada e non mercanteggiare su una tecnologia ormai obsoleta. A lungo termine, infatti, esisteranno, secondo Rubbia, soltanto due sorgenti di energia che permetteranno di abbassare la temperatura del pianeta e di risolvere anche i problemi dal punto di vista climatico: il solare nuovo e il nuovo nucleare. nucleare. Un nucleare capace di eliminare il problema delle scorie e di spezzare il rapporto malefico tra energia nucleare e usi militari, che punti sulla fissione fatta sul torio e non sull'uranio. Rubbia considera i reattori di terza generazione - ossia quelli per cui Berlusconi e Sarkozy hanno firmato il recentissimo accordo eccessivamente costosi e non meno pericolosi dei reattori di seconda generazione, i cui effetti abbiamo tutti visto e sentiamo sulla nostra pelle. Per un reattore di terza generazione occorrono dai 4 ai 5 miliardi di euro e per 4 centrali circa 14 miliardi di euro. il premio Nobel Rubbia aveva chiesto al Premier risorse per la sua ricerca sui nuovi reattori al torio. Per un reattore al torio, infatti, occorrono 500 milioni di euro, ossia una cifra ben meno esorbitante e più abbordabile.

La scelta di investire su una tecnologia superata e i cui punti critici riguardano scorie, approvvigionamento dell'uranio ed efficienza delle macchine (che sono ormai vecchie ed obsolete) non ci convince, così come ci lascia perplessi la strategia frettolosa e poco riflessiva di questo Governo. Se si vuole investire sullo sviluppo - e naturalmente l'asse portante dello sviluppo è l'energia - bisogna investire sul serio sulla ricerca. A differenza degli Stati Uniti, dove Obama sta investendo

profonda. Per quanto ci riguarda, la ricerca nel nostro Paese viene quindi ibernata. Mentre il mondo continua ad avanzare, noi firmiamo un accordo fuori dal tempo e portiamo avanti un disegno di legge che non può essere condiviso perché non va nel senso giusto con il giusto ritmo di marcia. Il provvedimento non convince soprattutto perché non dà garanzie e certezze all'intera comunità nazionale e allo sviluppo energetico del Paese, di cui si privilegia soltanto una una parentesi che altri Paesi stanno già superando e vogliono superare investendo quattrini nella ricerca scientifica e tecnologia (cosa che noi non vogliamo, né sappiamo fare). Da questo punto di vista,

infatti di puntare almeno sugli elementi base di una sicurezza da cui non si può prescindere e che invece il Governo sottovaluta pesantemente, con conseguenze che potranno essere veramente nefaste.

il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare. delega altresì il Governo alla definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate. Questa delega che viene data al Governo - dal nostro punto di vista, in bianco - ci preoccupa moltissimo, essendo la materia assolutamente delicata. Ecco perché il primo dei nostri emendamenti prevede la soppressione dell'articolo 14. Declinando poi altre formulazioni dell'articolo stesso, chiediamo che vengano comunque apportate alcune modifiche, che citerò per sommi capi.

del comma 2 inserisce tra questi princìpi e criteri direttivi anche la previsione della possibilità di dichiarare i siti «aree di interesse strategico nazionale», quindi soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione. Questo per il Gruppo dell'Italia dei Valori è in buona sostanza una sorta di militarizzazione del territorio. A questo proposito ci pare utile ricordare e rilevare che la popolazione italiana andrebbe convinta e non minacciata quando si devono assumere decisioni così importanti per un territorio. Quindi,

possa sostituirsi agli enti locali - questo pericolo è concreto - in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese. Esercitare i poteri sostitutivi e procedere di fatto al commissariamento degli enti territoriali interessati dalla scelta nucleare non ci sembra la strada migliore. Con l'emendamento 14.39 chiediamo che la prevista intesa con la Conferenza unificata debba comprendere non soltanto la costruzione e l'esercizio degli impianti, così come adesso prevede la norma, ma anche, ovviamente ancor prima, la loro localizzazione. In ultimo, con l'emendamento 14.43 chiediamo che al comma 2, lettera *g)*, dopo le parole: "autorizzazione unica rilasciata" vengano aggiunte le altre: «dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente». Questo perché la lettera *g)* introduce un principio delegato

siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con questo emendamento il Gruppo dell'Italia dei Valori invece intende subordinare la validità della suddetta autorizzazione all'ottemperanza delle procedure VIA e VAS previste dalla normativa vigente, procedure che rappresentano uno strumento per conseguire complessivamente elevati livelli di tutela e di qualità dell'ambiente.

Grazie,

oltre che alla Provincia e al Comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai Comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale,

a patto però che si ricomprenda anche l'ultimo periodo. Infatti è ragionevole escludere l'ultima parte dell'emendamento ove riferita all'intera legge, ma sarebbe oltremodo riduttivo se venisse eliminata quella previsione quando la stessa si riferisce esclusivamente al presente articolo. Quindi, chiedo al relatore e al rappresentante del la riformulazione, partendo dal presupposto che si accetta la limitazione al presente articolo e ovviamente la modifica della data che dovrebbe decorrere non già dall'assegnazione, ma dalla trasmissione degli schemi

tenuto conto delle limitazioni d'uso del territorio»; in altre parole, quella facoltà deve essere esercitata in ragione di uno specifico apprezzamento

Non ripeterò tutte le argomentazioni che avevo svolto in discussione generale, però mi permetto di ricordare che, oltre al voto fortemente contrario espresso dalla popolazione nel 1987 con il *referendum* in cui l'80,6 per cento dei votanti si era espresso contro la costruzione di centrali nucleari, ci sono argomentazioni fortissime che dovevano fare pensare il Governo e chi lo consiglia.

e costosa, non risolve il problema della dipendenza ed è poco responsabile verso le generazioni il motivo per cui è pericolosa: anche gli impianti più progrediti non garantiscono la piena sicurezza dal punto di vista tecnico, lasciando sempre un certo margine di rischio. Permettetemi: in uno Stato in cui crollano le case e i tetti delle scuole per mancata sicurezza, a maggior ragione posso esprimere questa preoccupazione

Inoltre, centrali nucleari sarebbero bersagli troppo convenienti anche per attacchi terroristici e - speriamo mai - bellici. Ho detto anche che è una scelta costosa. Ricordo che le ultime centrali di terza generazione costruite sono quella finlandese di Olkiluoto e quella francese di Flamanville, che invece

ma la dipendenza rimane, perché l'Italia non produce, non ha riserve di uranio e lo dovrà importare da quei pochi Paesi che lo producono, come l'Australia e il Kazakistan. abbiamo una grande dipendenza da questi Paesi. Oltre a questo, le organizzazioni internazionali ci insegnano che le attuali riserve di uranio dureranno

Sarebbe molto più responsabile se il Governo e chi lo consiglia - ripeto anche questo - puntasse sulle vie più moderne

Per non perdermi troppo nei dettagli, mi soffermo soprattutto sul risparmio energetico che è l'elemento più decisivo che può incidere sulla politica economica. Ho ricordato l'esempio della Provincia di Bolzano che punta, come la Germania e gli Stati Uniti di Barack Obama, al rilancio dei settori dell'energia rinnovabile (pannelli solari, energia eolica e termica), ma soprattutto alla casa clima.

l'articolo 14 delega il Governo ad emanare decreti legislativi volti a reintrodurre nel nostro Paese il nucleare, attraverso decreti che creeranno un sistema di norme per l'individuazione e la localizzazione degli impianti, degli stoccaggi

Noi proponiamo di sostituire la mera acquisizione del parere con un'intesa tra Governo e Conferenza unificata. Questo tipo di emendamento allevierebbe una delle critiche che non solo l'opposizione, il Partito Democratico, ma molta parte del Paese - che è attento a tali temi - ha rivolto in queste settimane a questo eccesso di centralismo.

che su una materia così delicata non si coinvolgano pienamente le Regioni. L'appello al Governo e al relatore è diretto anche a far comprendere che, su una tematica così complessa e delicata,

il parere negativo e ad accogliere il nostro emendamento.

Sottosegretario, mi permetto di insistere anche perché questa circostanza è riferita esclusivamente all'eventualità

su una materia e solo per questo articolo, mi permetto di insistere perché il testo venga approvato con questa specifica previsione.

di competenza e di esperienza in questo settore piuttosto variegato. Si intende dunque far valere quelle autorizzazioni e quelle validazioni concesse anche 10 anni fa nel nostro Paese, e ciò ci sembra eccessivo e non in linea con un Paese moderno, che ha a disposizione competenze, conoscenze e strutture in grado di vagliare le diverse opzioni tecnologiche in relazione agli interessi concernenti la sicurezza e la tutela

abbiamo presentato l'emendamento 14.306 perché consideriamo assolutamente rilevante la partecipazione dei cittadini ad un processo conoscitivo, se non decisionale, importante

tratta. Anche le direttive comunitarie vanno nel senso di allargare la base delle conoscenze sulle problematiche ambientali; ci meraviglia

Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori a questo ordine del giorno in quanto

le misure e le azioni che si intendessero assumere rispetto allo stoccaggio dei rifiuti nucleari vecchi e nuovi che si andranno a produrre, il Ministro ha dato una risposta molto laconica dicendo che effettivamente il problema

Presidente, al di là del merito estremamente importante di questo ordine del giorno, devo esprimere lo sconcerto del mio Gruppo: inizialmente infatti avevamo presentato un altro testo,

un modo di procedere che non può che lasciarci perplessi e veramente sconfortati rispetto a quello che ci lasciava supporre un lavoro di dialogo e di costruzione di un consenso con la maggioranza.

è la questione delle scorie nucleari e della compatibilità ambientale dei siti dove vengono stoccate temporaneamente e/o definitivamente è di estrema rilevanza e va ben al di là del riferimento al del riferimento al territorio del comune di Saluggia, dove uno di questi siti di stoccaggio è stato identificato. Se su una questione rispetto alla quale si era arrivati ad un accordo il parere del Governo è questo, immagino sul problema più generale dello stoccaggio temporaneo e/o definitivo delle scorie nucleari cosa mai potrà accadere nel dibattito che seguirà. Confermo comunque il voto favorevole del mio Gruppo.

Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime un voto contrario all'opzione proposta dal Governo in materia di realizzazione di centrali nucleari sul territorio nazionale. Le motivazioni di tale contrarietà non sono affatto di natura ideologica: la nostra è una contestazione di merito rispetto alle scelte e alle conseguenti implicazioni economiche. L'impostazione scelta dal Governo, come formulata anche nei recenti accordi tra Italia e Francia, porta benefici esclusivamente al sistema di imprese legate al nucleare francese. Le realizzazione delle centrali in Italia verrebbe affidata, anche dopo procedura di gara, ad imprese francesi che hanno le licenze e l'avanguardia tecnologica sul tipo delle centrali scelte e la nostra industria nucleare, quel poco che ne è rimasto, non verrebbe per niente coinvolta. Ovviamente l'ENEL ha fatto la scelta strategica probabilmente migliore per l'azienda sulla base dei suoi interessi, ovvero quella di sfruttare il legame che ha già da tempo con EDF, che è *leader* nel mondo nel nucleare. Rientrare nel nucleare dopo 20 anni di assenza, con un investimento che avrà un ordine minimo di 20 miliardi e senza avere dietro un progetto industriale rappresenta però un rischio economico assurdo. La dimensione dell'intervento impone di fare scelte che privilegino sistemi di ricerca, tecnologie ed imprese italiane, altrimenti il Paese avrà ridotto sì la dipendenza da gas, ma non quella dall'estero, che anzi si aggraverà. Il principale costo dell'uscita dal nucleare nel 1987 fu l'eliminazione dell'industria italiana nucleare, con alle spalle una lunga tradizione di ricerca e di avanguardia tecnologiche, che risaliva a Enrico Fermi. Se non si sfrutta l'occasione per riattivare il nucleare italiano, allora sarà un totale spreco, la cui ripercussione negativa è di portata strategica per il nostro Paese. Infatti, è poco verosimile, come si sostiene, che si possano fare gare per varie centrali nucleari e che queste non vengano vinte tutte dai francesi. Certo, alcune parti delle centrali, come quelle in cemento o gli acciai, potranno essere essere realizzate da nostre imprese, ma il grande valore aggiunto sarà nelle tecnologie, e queste, allo stato attuale, sono prevalentemente francesi. I Paesi che stanno investendo nel nucleare sono quelli che non possono uscirne. Il caso emblematico è quello della Gran Bretagna, che nel 2001 decise di chiudere le sue centrali, ma la messa in sicurezza veniva a costare 90 miliardi di sterline e divenne quindi obbligatoria la scelta di tenerle aperte e di cominciare a pensare ad ammodernarle. In tutto il mondo è difficile fare nuove centrali nucleari, in quanto si è scelto di andare verso assetti di mercato - su questo aspetto vorrei l'attenzione dei colleghi - dove gli ex monopolisti sono stati privatizzati e dove lo Stato si è disimpegnato da tali attività. Da allora è diventato difficile fare investimenti nel nucleare, perché nessun monopolista privato, mancando le garanzie dello Stato, è in condizione di garantirsi ricavi certi da questo tipo di intervento. - non arriverebbero benefici da un supposto minor costo dell'energia da nucleare, perché l'investimento sul nucleare trova la propria ragione essenziale se serve a sviluppare un sistema di imprese ad alta tecnologia, esattamente come hanno fatto i francesi, che esportano licenze, tecnologia e *know-how*. Pensare di investire molti miliardi di euro solo per ridurre il costo di produzione non ha adesso un senso economico. Tale costo non verrebbe affatto ridotto: è difficile sostenere che il nucleare, allo stato attuale e nel medio e lungo termine, possa avere enormi vantaggi economici rispetto al ciclo combinato a gas, che noi abbiamo in abbondanza. Il sistema elettrico italiano ha un eccesso di capacità di proporzioni storiche e non capisco perché non lo si dica. Le statistiche di TERNA parlano di una capacità elettrica di oltre 90.000 MW, con una punta di domanda che in Italia è stata raggiunta solo nel 2007 con 60.000 MW. nuove centrali nella pianura padana sono utilizzate a meno del 50 per cento del loro potenziale. Pensare di fare nuove centrali in Italia in questo momento è un paradosso economico e rappresenterebbe un ulteriore costo che finirebbe sui già alti prezzi dell'energia. Le nuove centrali realizzate negli ultimi 10 anni sono soprattutto cicli combinati a gas per quasi 30.000 MW. In Europa nessun Paese ha realizzato tanta capacità elettrica

È vero che siamo troppo dipendenti dal gas importato, ma il problema, al punto in cui siamo, va risolto diversificando gli arrivi di gas, ovvero facendo finalmente i rigassificatori. Un eventuale rientro nel nucleare presuppone un chiaro indirizzo di politica industriale ed energetica, definita e condivisa in Parlamento, aperta al confronto con le Regioni e con le comunità territoriali. Tale politica non c'è: fa ancora testo il Piano energetico nazionale del 1988. Le cinque centrali previste utilizzerebbero la tecnologia EPR, che prevede una dimensione grande, di 1600 MW per centrale, che richiederebbe quantità d'acqua tali da escludere tutte le localizzazioni sul Po. Si dovrebbe andare sul mare, lungo le coste, e vi sarebbero enormi resistenze a quell'insediamento e un grande costo nel convincimento delle popolazioni, che non si può bypassare attraverso la definizione di "area di interesse strategico nazionale".

- non solo e non tanto per problemi legati alla maggiore sicurezza, quanto piuttosto perché utilizzano le scorie e riducono l'impiego di uranio, le cui riserve scarseggiano. Quelle di quarta generazione utilizzano scorie di precedenti centrali o altre scorie, e le disponibilità sono molto più abbondanti.

Ma per l'Italia la cosa più importante è che per queste centrali si può sfruttare la ricerca già avviata in passato dall'Enea e sviluppare licenze industriali italiane esportabili in Paesi in Paesi come la Cina e l'India, nei quali si giocherà in futuro la *leadership* di questa fonte energetica, che ha il grande pregio di non emettere CO2. Per queste considerazioni, che, come vedete, non propongono una lettura antinuclearista,

ma anche la nostra disponibilità, qualora ve ne fossero le condizioni, anche di praticabilità democratica, a concorrere alla definizione di una nuova e più avveduta politica energetica nazionale, coerente con gli ordinamenti comunitari e le più moderne visioni internazionali. *(Applausi

Grazie,

Non comprendiamo il motivo di un prelievo dalla componente A2 in bolletta e della relativa destinazione a bilancio, dato che non è giustificata da un opportuno impiego per ridurre gli oneri A2 dell'attività di *decommissioning* e che tale misura graverà comunque in bolletta a carico di consumatori e utenti.

Mi richiamo ai motivi ben espressi dal senatore Sangalli nella sua dichiarazione di voto sull'articolo 14, che hanno evidenziato con forza quanto sia necessaria una sede democratica di discussione su un argomento così delicato come l'energia nucleare. Con questo emendamento si propone di istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di confronto in materia di energia nucleare per discutere le proposte economiche e tecniche, soprattutto il dettaglio dei costi degli investimenti, oltre che i tempi di realizzazione e gli effetti della ripresa di una produzione di energia nucleare. A questo tavolo dovrebbero partecipare le maggiori organizzazioni nazionali delle parti economiche e sociali rappresentate nel CNEL oltre che i rappresentanti del del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nell'ambito dell'introduzione dell'energia nucleare nel nostro Paese, si ritiene assolutamente necessario intavolare un costruttivo dibattito su una politica energetica di ampio respiro e dai contenuti strategici, non soltanto collegati alla contingenza dei provvedimenti di legge emanati. Considerata la delicatezza e la complessità del problema di un nuovo piano di sviluppo del nucleare dal punto di vista anche socio-ambientale, il tema deve essere affrontato

dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva.** *(v.

irrispettoso nei confronti delle istituzioni.

Senatrice Incostante, la senatrice Segretario Amati sta verificando. Chiedo ai colleghi senatori di ritirare le schede dei colleghi assenti.

Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico. Con l'articolo 15 si affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare: ci pare veramente eccessivo. Sarebbe stato molto più saggio approdare ad una scelta così importante dopo aver operato una specifica ricognizione e una valutazione degli impianti e delle tecnologie presenti sullo scenario internazionale, dei relativi costi di realizzazione e di gestione, della frequenza di casi di malfunzionamento o di incidenti verificatisi nel corso dell'esercizio relativamente alle diverse tipologie di impianti. Per questo voteremo contro l'articolo

Colleghi, per cortesia, ci sono i senatori Segretari che verificano. Portate pazienza, è inutile urlare da una parte all'altra: "La scheda! Togliete la scheda". Senatrice Amati, prego;

nella votazione n. 24 risulta aver votato - non me ne voglia - il senatore Comincioli (che non vedo già più), che è entrato successivamente. Inoltre, nella

Per cortesia, senatore Legnini e senatrice Incostante! Ho chiesto ai senatori Segretari di far ritirare le schede in più. Mi sembra che questa Presidenza stia dando attuazione alle regole che ci siamo dati. Metto

come è stato formulato, porti ad un vero e proprio smantellamento della Sogin, che, sappiamo tutti, ha un'esperienza pluriennale nell'ambito della gestione dei rifiuti radioattivi.

con il quale chiediamo che la partecipazione dello Stato in altre società operanti in questo delicatissimo settore sia almeno del 40 per cento e non del 20, così come proposto all'Assemblea. Il successivo emendamento 16.110 di fatto è volto ad evitare l'estromissione delle Regioni dalle procedure di valutazione d'impatto ambientale e di autorizzazione alla perforazione per la ricerca di idrocarburi. Abbiamo visto che in questo provvedimento troppo spesso si tende a togliere qualsiasi potere (e quindi qualsiasi potere decisionale) alle Regioni e agli enti locali. In particolare, nel comma 19 dell'articolo 16 si va appunto nella direzione di estromettere le Regioni. La valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione per la perforazione vengono affidate, così com'è formulato il comma 19, all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, competente a seguito di un non meglio precisato procedimento unico, al quale partecipano la Regione e gli enti locali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità della legge n. 241 del 1990. Questo significa, a nostro parere, che la volontà delle Regioni possa essere in questi casi totalmente scavalcata dallo Stato, oltretutto andando assolutamente in senso contrario ad una politica di federalismo che lasci ai territori le scelte decisionali, soprattutto quando si tratta di scelte così importanti. L'emendamento 16.110, volto appunto a sopprimere il comma 19, va nella direzione che ho

In modo molto solerte, i Comuni delle isole minori hanno redatto un Documento unico di programmazione delle isole minori (il cosiddetto DUPIM) ed hanno indicato i progetti che si possono realizzare immediatamente

2008 hanno inoltrato i suddetti documenti al Dipartimento per gli affari regionali, come sancito dalla legge finanziaria, corredati dalle delibere dei Comuni e delle Regioni attestanti la coerenza della programmazione comunale con quella regionale e indicanti i progetti DUPIM che sarebbero stati finanziati dalla Regione, nonché gli altri interventi che sarebbero stati ulteriormente finanziati perché correlati allo sviluppo delle aree comunali.

unificata, come previsto dalla finanziaria 2008. Con le relative erogazioni del Fondo i Comuni erano pronti ad aprire i cantieri. Anzi, voglio ricordare ai colleghi - e so che molti di voi hanno a cuore il problema delle isole minori che fanno parte delle vostre Regioni

perché con esso il Governo cambia radicalmente la procedura prevista dalla finanziaria 2007, confermata nel 2008, per l'assegnazione del Fondo di sviluppo delle isole minori,

i Comuni delle isole minori, riuniti nell'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori, hanno elaborato un Documento unico di programmazione e, attraverso esso, indicato i progetti da realizzare immediatamente (dunque, le priorità a medio e breve termine); concordemente hanno individuato i criteri di riparto,

Grazie, Con la relativa erogazione del Fondo i Comuni erano pronti ad aprire i cantieri; anzi, in alcuni casi questi sono stati avviati poiché l'adempimento statale finale avrebbe già dovuto essere approvato considerando che sono passati oltre quattro mesi. Non si capisce dunque come si possa spiegare agli oltre 200.000 abitanti delle isole minori, ai 37 Comuni e alle 7 Regioni interessate che il lavoro concluso deve ricominciare. Pensiamo che la volontà di far partire l'economia non si consegue fermando i cantieri. Quindi la formulazione del comma 9 dell'articolo 16 risulta veramente incomprensibile. pertanto che essa venga modificata, che i criteri e le priorità siano decise dall'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori, di concerto con i Ministri interessati, e che con il decreto proposto dal Ministro per gli affari regionali vengano individuati gli interventi ammessi al finanziamento. **Saluto

l'emendamento 16.76 propone che la facoltà, concessa ai Comuni, di destinare le aree in loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e alla produzione, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici,

dei propri soci il beneficio che ricevono dall'accesso a tale facoltà. Credo che sia assolutamente evidente l'impatto positivo che l'estensione della norma avrebbe rispetto allo scopo dell'articolo, che è quello di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili, in relazione alla grande estensione delle attività della cooperazione di abitazione, che nel nostro Paese ha realizzato, ad oggi, oltre 900.000 abitazioni, contando quindi quasi un milione di soci.

su una riformulazione

mi rimetto al Governo, che credo chiederà una riformulazione.

e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente». Inoltre, al punto *c)*, sempre in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione bilancio, dove è scritto «individuare i criteri per determinare», viene aggiunto «senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica».

Colleghi, per cortesia,

sui commi 6 e 7 che, come noto, puntano a modificare l'assetto societario della Sogin spa e a commissariarne il consiglio d'amministrazione. Questa società, che si occupa peraltro del cosiddetto *decommissioning* in materia di impianti nucleari, ha una sua specificità professionale. È una società interamente partecipata dallo Stato e ha una missione molto delicata in tema di energia nucleare.

Ciò consentirebbe l'ingresso, che può essere legittimo, di altre società private che hanno una competenza specifica nel settore, ma

In questo contesto non si spiega neanche il motivo per il quale si debba procedere alla nomina di uno o più commissari per la gestione della Sogin,

queste norme non assicurano alcunché sotto il profilo del futuro dei lavoratori impiegati in questi settori, che si occupano in maniera professionale di un'attività così delicata. E sinceramente nel quadro strategico del rilancio del nucleare - su cui siamo d'accordo - non comprendiamo le ragioni per le quali si debba procedere con la privatizzazione della Sogin e con il suo commissariamento,

cioè un rilancio degli studi, della ricerca e dell'attività nel settore dell'approvvigionamento energetico da fonte nucleare. Non comprendiamo perché debba essere smantellata questa società che si occupa in maniera professionale di un'attività delicata e perché si debba compromettere il futuro di lavoratori che non sono peraltro facilmente reimpiegabili, perché si trovano in quel una vita e perché da quando questa società è nata si occupano di questi problemi, si dedicano solo ed esclusivamente della sicurezza dello smantellamento delle centrali nucleari. delle centrali nucleari. Crediamo sia opportuno che questi due commi vengano espunti dal testo, perché riteniamo possano essere nocivi e pericolosi rispetto alle strategie che ci siamo, o che vi siete, prefissati.

al fine di operare il doveroso approfondimento, con il quale sarebbe opportuno chiarire molti aspetti: non solo relativamente alla norma, che non appare chiarita, circa le procedure per il commissariamento di una società (che non presenta elementi propri di un intervento di commissariamento), ma per le questioni legate alla sicurezza nucleare nel nostro Paese e all'attività di *decommissioning* che la Sogin sta finalmente realizzando con efficacia e efficienza.

riferita all'oggetto del piano che il Ministero dello sviluppo economico redige ogni anno in relazione al piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico.

Grazie, la collega stava svolgendo il suo lavoro, perché ritengo che se certe disposizioni sono date dalla Presidenza, esse valgono per la parte di destra dell'emiciclo e per quella di sinistra. Tuttavia la collega è stata respinta dalle

*(PD)*. Mi dispiace intanto dover dire al presidente Quagliariello,

è essenziale che il controllo sia fatto in modo rigoroso. Vorrei però aggiungere qualcos'altro: un paio di mesi fa, primo firmatario il senatore Livi Bacci,

Dichiaro aperta la votazione.

principi vincolanti da rispettare in maniera acritica, ma introducono semplicemente una modalità di intervento tesa a mettere in campo lo sforzo che è necessario produrre per garantire migliori condizioni di sicurezza, migliori condizioni di tutela della salute, migliori condizioni di rispetto dell'ambiente. Tali obiettivi sono tutti conseguibili

nella condizione di impiegare. Anzi, proprio questo approccio rende più competitivi i nostri operatori,

rinunciare ad esercitare un'azione di stimolo per l'innovazione tecnologica, per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili a tutela della salute dei cittadini e della qualità ambientale ci sembra una posizione non comprensibile. Si rinuncia a mettere in campo un'azione che non solo può rendere il nostro Paese ancora più protagonista sul sul versante interno, ma che può anche incrementarne la capacità competitiva a livello internazionale. l'utilizzo di queste metodologie determina anche condizioni utili per ottenere il consenso delle popolazioni interessate, per realizzare la necessaria condivisione da parte degli enti locali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Per questo motivo, rivolgo un appello a rivedere il parere contrario e ad accettare questa impostazione, che risponde - ripeto - agli interessi del nostro Paese.

senatori Bubbico, Chiurazzi e ad altri colleghi, relativo alla situazione di crisi che sta interessando il distretto del mobile imbottito dell'area murgiana, che sta portando alla progressiva perdita di quote di mercato interno ed internazionale, alla riduzione del numero delle imprese e alla perdita di numerosi posti di lavoro. Considerando l'urgenza della crisi produttiva, che incrocia una crisi sociale devastante per migliaia di famiglie, si chiede che il Governo venga in Aula a riferire con urgenza, per conoscere se e quali provvedimenti immediati intende adottare a sostegno del distretto del mobile imbottito dell'area murgiana.

al sottosegretario con delega al turismo Michela Brambilla, nel quale si chiedono chiarimenti in merito all'attuazione dei buoni vacanza. A tutt'oggi non ho ricevuto risposta: le aspettative che si sono create a seguito di questo provvedimento sono enormi, ma non sono ancora stati forniti chiarimenti sull'attuazione.

gli obbligazionisti di titoli Lehman Brothers, i quali sono nostri concittadini che rischiano di essere i soli risparmiatori privi in questo Paese di qualunque tutela. La richiesta è stata formulata per conoscere da parte Grazie,

Presidente, desidero sollecitare il Governo a seguire la vicenda della FIAT di Termini Imerese, in Sicilia, e anche a riferire in Aula non appena sarà opportuno e possibile.

che guardi all'espansione del settore dell'automobile nel Mediterraneo e in particolare nei Paesi del Nord Africa. Si potrebbe pensare, quindi, alla possibilità di produrre lì innovazione e di creare anche un'opportunità senza precedenti,

che il Governo intervenga, sia attivo, sia in grado di immettere anche in questa valutazione delle risorse e venga qui a riferire appena - ripeto - le condizioni lo detteranno. Senatore Lumia, sarà mia cura informare il presidente Schifani dell'osservazione da lei svolta nel suo intervento e sollecitare il Governo.

in relazione al terremoto nella Regione Abruzzo, ma i Vigili del fuoco da anni si battono per essere riconosciuti in funzione di quella attività espletata, che è poliforme, e hanno avuto un'alta percentuale di morti e malattie professionali causate dall'espletamento della loro missione in favore della tutela e della sicurezza dei cittadini che si possono ricomprendere nel novero di quelle categorie usuranti. Quindi, al di là degli elogi che vengono fatti dal Governo alle forze dell'ordine e a tutto il settore del comparto del volontariato che riguarda la sicurezza, noi dobbiamo al Corpo dei Vigili del fuoco una risposta. Il silenzio assordante del Ministro dell'interno da luglio ad oggi nel fornire una risposta doverosa nei confronti di una rivendicazione che da anni viene portata avanti in relazione a mansioni effettivamente espletate, anche con il rischio di incolumità personale e con grande generosità, ci sembra un fatto strano, considerata anche la